delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, i subemendamenti 2.100/1, 2.100/2 limitatamente alla seconda parte e 4.100/2, in quanto non direttamente correlati agli emendamenti ai quali si riferiscono.

*(PD)*. Signora Presidente, vorrei scusarmi con tutti i colleghi per questa attesa e per il fatto che i nostri lavori cominciano con un po' di ritardo. Al tempo stesso, però, credo che il lavoro svolto dai colleghi della Commissione bilancio meriti queste parole. Se abbiamo fatto attendere l'Assemblea ieri pomeriggio e questa mattina è perché sono arrivati in zona Cesarini un certo numero di emendamenti dei relatori corredati opportuni subemendamenti che hanno imposto alla Commissione bilancio un supplemento di lavoro. Preciso questo affinché sia chiaro non abbiamo interrotto i nostri lavori pomeridiani di ieri perché la Commissione bilancio non aveva fatto il suo lavoro; la Commissione bilancio ha dovuto fare un'altra parte di lavoro perché sono pervenuti nuovi emendamenti e subemendamenti da esaminare. Come voi sapete, ciò impone un'istruttoria tecnica da parte dei nostri Uffici, che voglio qui ringraziare perché si sottopongono sempre a ritmi davvero estremi,

dall'articolo 81 della Costituzione, che è uno dei pilastri fondamentali del nostro lavoro. Dico questo per due ragioni. La prima è perché resti a verbale l'esatto svolgimento degli avvenimenti di queste ore. La seconda, per un appello a tutti i colleghi. Dato che stiamo andando verso una fase concitata della nostra attività, perché prima dell'interruzione estiva, come sempre, si accumulano tante questioni, se le Commissioni riuscissero a concludere in maniera netta il loro lavoro, senza code che comportano un allungamento dei tempi, questo ci aiuterebbe ad essere efficienti e a produrre in modo ottimale le decisioni che l'Assemblea è chiamata a prendere. si faccia un lavoro il più ordinato possibile: consegnate alla Commissione bilancio il lavoro una volta concluso, in modo da poter espletare tutte le procedure che ci competono una volta sola e non più volte, creando indubbi

sono volti ad affermare la posizione del nostro Gruppo rispetto alle missioni internazionali ma, soprattutto, al modello di difesa che vorremmo si affermasse. Abbiamo chiesto in Commissione difesa, proprio quest'anno, l'avvio di un'indagine conoscitiva per indagare nel dettaglio i risultati raggiunti nelle missioni internazionali in cui l'Italia viene impegnata ma, soprattutto, per verificare e, se possibile, interpretare una difesa differente e sostenibile, come noi la definiamo. Dalle audizioni in Commissione di organizzazioni non governative, come Amnesty International, sono emersi dati importantissimi che potrebbero rivoluzionare il modello di difesa tradizionale,

di migranti, cioè a combattere il traffico illecito di esseri umani. Noi vorremmo continuare a insistere, perché fare la lotta al traffico illegale significa anche stroncare vie di finanziamento al terrorismo. Abbiamo visto, infatti, che tutti i soldi pagati da quei disperati finiscono nelle casse delle organizzazioni parallele e legate alle organizzazioni di terrorismo internazionale.

finiremmo per dare solo il messaggio che è molto semplice arrivare nel nostro Paese; alimenteremmo le speranze; alimenteremmo il numero di persone stimolate a partire; alimenteremmo le casse del terrorismo internazionale.

il più grande problema che affronta oggi la comunità internazionale è proprio il contrasto al terrorismo internazionale. Ieri è toccato alla Turchia, giorni addietro è toccato alla Nigeria, alla Tunisia, all'Egitto, alla Libia e via dicendo. In Europa è toccato al Belgio e alla Francia. Per fortuna

che queste missioni devono servire a contrastare il terrorismo e non a fare semplificazione dei traffici verso il nostro Paese, perché questo vuol dire stimolarne altri e sempre più e arricchire le casse del terrorismo internazionale.

sui temi dell'immigrazione, che sono una causa non secondaria della crisi dell'istituzione europea, dell'esito del*referendum* britannico e della pressione dei popoli, molto critici nei confronti di un'Europa che non sa gestire i temi dell'immigrazione. Quindi, governarli in maniera demagogica può portare a una dissoluzione dell'Unione. Siccome di Europa ne abbiamo una, cerchiamo di non sfasciarla con gli interrogativi

Avete mai visto dei rimpatri? Ieri il Ministro dell'interno ci ha ricordato che sono stati espulsi 95 soggetti, che non sono clandestini, ma sono considerati potenziali terroristi. Ma, per quanto riguarda l'espulsione dei clandestini che non sono terroristi, le cifre credo siano pari a zero. Per quanto riguarda la ricollocazione dei profughi all'interno dell'Europa,

comporta che tante navi circolino nel Mediterraneo e, siccome gli scafisti lo sanno, organizzano le partenze dei clandestini sapendo che, dopo poche miglia, la nave tedesca, italiana o francese li soccorrerà e li porterà in Italia.

è talmente vero che si può fare il conto alla rovescia non di quanti sono pronti a partire ma di quanti ne arrivano in Italia. In quattro giorni sono 12.000. Altro che 300.000 nel giro di alcune settimane!

bene a non coltivare simili illusioni. Ma una politica di sicurezza e di solidarietà ha delle scadenze, dei tempi e, quindi, anche l'operazione EUNAVFOR MED non può continuare all'infinito se la fase 3, di vera lotta allo scafismo nelle acque libiche, non scatta. Si dice: signori, noi ci fermiamo, e poi qualche soccorso ci sarà lo stesso; ma noi oggi abbiamo moltiplicato

o quella guerra fondamentalista che anche in Libia, e non solo negli aeroporti di Bruxelles, di Istanbul o di altri luoghi, si manifesta con le sue deflagranti e tragiche situazioni. Questo provvedimento sulle missioni internazionali, quindi, cari colleghi,

costiera e ciò rappresenta uno sviluppo importante. Certamente la missione EUNAVFOR MED - come si è detto più volte - tende all'obiettivo di arrivare alla terza fase per raggiungere le coste libiche, ma la strategia condivisa unanimemente, per non commettere gli errori del passato, è soprattutto di andare d'accordo con la

ha raggiunto importanti obiettivi: diverse centinaia di imbarcazioni non sono più utilizzate dagli scafisti la capacità operativa degli stessi è stata molto ridotta. Certamente dobbiamo arrivare ad una terza fase. Ne approfitto, poiché proprio in questi giorni è cambiato il comando della missione, per salutare l'ammiraglio

la domanda è retorica perché non può avere risposta. Sappiamo quando potrà scattare la fase 3, quella in cui il Governo Serraj della Libia potrà chiederci di agire anche nelle acque libiche per contrastare l'attività degli scafisti? Non lo sappiamo, perché siamo al corrente, colleghi, che in Libia è ancora in corso uno scontro che noi ci auguriamo - e su questo la pensiamo come il Governo - premi l'azione del Governo Serraj e si possa assumere un controllo reale del territorio. Tuttavia, tra la presenza perdurante di gruppi fondamentalisti che controllano pezzi di territorio, il contrasto con Haftar

Quindi, noi abbiamo una data incerta. Abbiamo sollevato il problema più volte, anche nella precedente conversione di decreti, l'abbiamo sollevato in tutte le discussioni riguardanti i vertici europei. Ho appena ricordato che la nostra risoluzione, accolta dal Governo lunedì,

più di altre, nel votare il recente *referendum*, si è molto orientato all'immigrazione, pensando al modo con cui la politica europea fallisce. Renzi ci dice poi che ha proposto il *migration compact*, un grande programma in Africa. Dov'è? Non ne hanno parlato nemmeno ieri, frastornati dal risultato inglese. Non si è ancora capito quali siano le conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, se non che Juncker faceva gli scherzi a Farage o altre polemiche del genere. partecipare ad uno qualsiasi dei programmi televisivi e non c'è bisogno delle istituzioni. Noi chiediamo caldamente di votare a favore dell'emendamento 1.8 (testo 2), che pone una data limite a questa operazione che non sta raggiungendo le finalità che si è prefissa e di cui abbiamo discusso. Prima il relatore si complimentava con gli ammiragli che si alternano al comando di questa operazione.

Vedete la nemesi della storia: Cameron e Sarkozy, entusiasti della guerra libica alla quale costrinsero l'Italia, oggi annaspano o vengono sconfitti, forse anche per quegli errori strategici. Forse, infatti, l'Europa ha cominciato a distruggersi sbagliando tra amici e nemici, perché alcuni che erano cattivi amici forse erano utili

poi le ragioni della solidarietà e dell'accoglienza troveranno i modi fisiologici per esprimersi. Tuttavia, il modo di gestire questa vicenda è approssimativo e si scarica sull'Italia, perché la solidarietà europea non l'abbiamo vista. Altro che rivedere i trattati di Dublino sui profughi e sui clandestini, che portano con le navi, come ho già detto prima e non mi ripeto. Noi invitiamo, quindi, l'Assemblea

che ci siano grandi sviluppi. Non è un emendamento banale, ma rappresenta un'occasione per il Senato per inviare un segnale per una politica che abbini alla solidarietà il giusto realismo nella gestione della crisi mediterranea.

ampio. Ciò significa che la sensibilità su questo argomento è abbastanza diffusa, ancorché le logiche di partito obblighino a voti abbastanza serrati.

presso gli organismi internazionali affinché nei mandati delle missioni internazionali siano inseriti esplicitamente, ove pertinenti, gli obiettivi di protezione della popolazione civile». è favorevole inserendo nel dispositivo, dopo le parole: «a fornire al Parlamento», le parole: «nell'ambito delle previste comunicazioni rese dal Governo sulle missioni internazionali».

l'impegno rimane quello proposto, anche perché riteniamo che la genericità del medesimo dia comunque anche la possibilità di di coprire la parte giuridica e le sanzioni delle violazioni del principio di protezione del medesimo, tenuto conto che è assolutamente esplicitato che gli obiettivi degli organismi sono di protezione della popolazione civile.

e sta diventando cronica. Illustro contemporaneamente anche l'emendamento 2.5, che vorrebbe specificare che la missione in Afghanistan si conclude

arabi. Tanto varrebbe che andassimo direttamente noi, con le nostre Forze armate, a bombardare lo Yemen, dove anche ieri sono morte decine e decine di persone. Questa è l'attenzione

più che di interloquire con le forze libanesi. In più di un'occasione le nostre forze hanno intercettato convogli probabilmente trasportavano armi e si dedicavano a traffici illegali e l'unica cosa che hanno potuto fare è stata la segnalazione alle autorità libanesi.

con il mio ordine del giorno G2.100 voglio soffermarmi sui riferimenti alla Croce Rossa inclusi in questo provvedimento. Pur apprezzando l'atteggiamento che si intende riservare alla continuità operativa della Croce Rossa,

possa non essere uno strumento pienamente efficace. Tutto questo in ragione del fatto che si è inteso limitare, per quanto attiene al corpo militare, il coinvolgimento ai soli trecento di cui all'aliquota dedicata, lasciando fuori la restante componente del corpo, destinata quindi all'inesorabile smilitarizzazione. Purtroppo, sappiamo che questa struttura servirà da paracadute a quella attuale, consentendo anche una più agevole gestione delle risorse. Lo ribadisco: di opportunità e non di funzionalità. Ma si fa fatica a capire in che modo questo sistema, che prevede un complesso assemblaggio di personale, strutture ed altro possa garantire un efficace funzionamento. Pertanto, chiedo che comunque venga preso in considerazione l'impegno di cui al mio ordine del giorno G2.100, al fine di sospendere questa cosiddetta procedura di smilitarizzazione, anche alla luce di rinnovati e potenziali impieghi del personale del corpo militare della Croce Rossa, determinando eventuali soluzioni alternative per il coinvolgimento del corpo militare della Croce Rossa, valutando l'ipotesi, in ottemperanza agli impegni già accolti da Governo in più occasioni, di inquadrare l'operatività del corpo militare della Croce Rossa, nella sua totalità, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea, così come ribadito in molte altre occasioni dal Ministero della difesa.

una soluzione istituzionale, che poi è venuta con l'emendamento dei relatori. Quindi non abbiamo presentato emendamenti analoghi, proprio per semplificare i nostri lavori. Tuttavia l'ordine del giorno del senatore Di Biagio richiama una questione che diversi di noi in Parlamento hanno più volte sollevato, non ho mai capito quale sia poi la risposta vera del Governo. Mi riferisco alla smilitarizzazione-soppressione della Croce Rossa militare: è vero che c'è la sanità militare e che ci sono altre strutture, però, francamente,

con auto-danno del Governo, siamo comunque favorevoli all'impianto del decreto). Vorrei richiamare l'attenzione del sottosegretario Rossi, anche per le sue consolidate precedenti esperienze,

spesso è stata proprio la Croce Rossa militare ad aver dato un senso solidaristico a queste missioni, garantendo l'assistenza sanitaria non solo ai nostri militari, perché una volta realizzati dei presidi, questi sono stati utilizzati largamente dalle popolazioni locali.

e recepisca le istanze che questo ordine del giorno nuovamente sollecita e per questo ha la nostra condivisione non occasionale - come ben sa il senatore Di Biagio - ma operosa e costante. Il senatore Di Biagio ha avuto la tempestività di rinnovare questo ordine del giorno e noi ci associamo nella firma e nel voto.

«a valutare, in ottemperanza agli impegni già accolti dal Governo, di inquadrare l'operatività del Corpo militare croce rossa italiana nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea».

nell'obiettivo principale che è quello di trovare un'operatività al Corpo militare della Croce Rossa in prospettiva e soprattutto in funzione europea, che è l'ambito in cui

oneri aggiuntivi, trattandosi semplicemente di un presidio militare e specificandosi che questo presidio militare avrà anche il compito,

che così, in questi termini, inquadrerebbe oggettivamente l'esigenza operativa del corpo militare della Croce Rossa nella sua totalità nell'ambito dei meccanismi di protezione civile

di sostituire dal termine: «la sospensione» con le parole: «rivalutazione dei termini di smilitarizzazione al fine di garantire la continuità operativa del Corpo». ho già detto nel mio intervento, la smilitarizzazione è un tassello importante del processo di privatizzazione. O decidiamo che non facciamo più niente e chiudiamo la questione, oppure, se se decidiamo che la smilitarizzazione è un tassello importante, con gli strumenti che prevede la normativa vigente cerchiamo di gestire il problema. Non possiamo intervenire su questo punto. Questo è allo stato. Per fare altre cose dobbiamo

Poiché abbiamo discusso ripetutamente della necessità di avviare un percorso di distensione nei rapporti tra e Russia, queste due operazioni a noi sembrano molto provocatorie e non vanno sicuramente nella direzione di una distensione con la Russia, che è il Paese che più di ogni altro aiuta tutti i Paesi europei a lottare contro il terrorismo internazionale. [DI

ferroviario dichiarato fuori servizio. Preciso che da parte del Governo di Asmara vi è l'impegno, già più volte garantito, alla presa in carico delle spese logistiche di trasporto di questo materiale. Si continua a disattendere un impegno contratto ormai da quattro anni, legittimato da provvedimenti legislativi varati dal Parlamento e supportati dal Governo, osservando un accordo e animando la violazione di una sorta di legittimo affidamento da parte dell'Eritrea che porterebbe, allo stato attuale, a compromettere le già scarse relazioni tra i due Paesi. Pertanto l'Italia non può continuare a ignorare un impegno già assunto, soprattutto se già ratificato dal Parlamento, per ben due volte su iniziativa del Governo stesso. Per queste ragioni, chiedo al Governo di accogliere l'emendamento 4.4, per dare finalmente credibilità alle promesse fatte dal nostro Paese.

dal valore prettamente simbolico e politico e attiene alla cessione di materiali che l'articolo 4, comma 6, del provvedimento autorizza ad effettuare nell'anno 2016,

la Repubblica araba dell'Egitto, alla quale verrebbero donati una serie di pezzi di ricambio per gli F-16 che hanno in quel Paese. Il motivo di questo emendamento è ovviamente di fare pressione sul nostro Governo testimoniando, dopo le parole che in quest'Aula molto intensamente si sono sentite da tutte le parti politiche sulla vicenda

Non si tratta di un atto di ostilità rispetto alla Repubblica araba d'Egitto, che continua a essere un Paese nostro alleato e del quale riconosciamo anche il valore strategico in questo momento nella vicenda più complessa che riguarda la lotta al terrorismo; tuttavia riteniamo che il nostro Paese abbia titolo e diritto, come ha fatto quando ha richiamato l'ambasciatore e con numerosi atti successivi, a continuare a tenere sotto pressione Nella discussione generale su questo stesso argomento si sono dette cose che sono andate oltre alle intenzioni delle Commissioni quando hanno presentato questo emendamento. Le intenzioni sono di agire in modo politico su una questione che è prettamente simbolica, conferendo al nostro Governo la condizione per poter rapportarsi con la Repubblica araba d'Egitto in modo soggettivo. Altre soluzioni che abbiamo sentito nella discussione generale, che prevedono interventi drammatici, non fanno parte della filosofia di questo emendamento e del nostro indirizzo politico.

non l'ho capito.

L'emendamento risponde a una richiesta specifica da parte della Somali Police Force

PRESIDENTE. I pareri favorevoli sugli ordini del giorno sono relativi a delle riformulazioni, ma nessuno mi dice quali sono queste riformulazioni.

a rinnovare l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12 alla citata cessione nell'ambito fino alla fine. Questa parte viene sostituita con la seguente: «una volta verificato il perdurante interesse da parte eritrea alla cessione e conferma circa la disponibilità ad assumersi tutti i costi relativi alla raccolta e trasporto del materiale e tenendo conto dell'evoluzione del quadro politico interno eritreo anche sotto il profilo dei diritti umani e delle libertà fondamentali». Per l'ordine del giorno G4.101 la la riformulazione proposta è la seguente:

concernente la nostra partecipazione militare alle attività NATO di rassicurazione degli alleati baltici e polacchi, ritirandola o riducendola a livelli veramente simbolici; con le seguenti: «alla luce degli impegni militari assunti con ONU, Unione europea o NATO o prevedibili in altri scenari, a partire dal Mediterraneo».

con le seguenti: «si mantenga negli stretti limiti previsti dalla regole di ingaggio della missione NATO per la difesa del territorio e della popolazione della Turchia contro le minacce poste da possibili lanci missilistici oltre il confine siriano».

un alleato con il quale c'è una controversia riguardante la vicenda drammatica dell'uccisione di Regeni e non devo stare qui a descrivere

anni sta colpendo, tra l'altro, non solo alcuni obiettivi occidentali, quali l'aeroporto di Bruxelles, non solo probabilmente - non lo sappiamo ancora, siamo qui in Aula - da quello che dicono le autorità turche, l'aeroporto di Istanbul, ma ha colpito il turismo

forse - viaggerà di meno verso il Nord Europa. Del resto, se diciamo che bisogna contenere l'immigrazione, allora bisogna anche aiutare lo sviluppo. Che c'entra questo? Ricordo che in Egitto il terrorismo colpisce anche obiettivi egiziani

Al-Sisi è un militare e, quindi, vi è una sorta di continuità. Rotto il legame con i russi, gli americani sono diventati i grandi *sponsor* dell'Egitto, considerato un baluardo nei confronti del fondamentalismo e anche una realtà che poi, con Israele e altri Paesi, è passata a siglare trattati e accordi che costarono la vita

ai colleghi - stiamo votando un atto di ostilità all'Egitto dicendo: non vi diamo i pezzi di ricambio degli aerei che vengono usati anche in Libia per contrastare i fondamentalisti che occupano Sirte e altri luoghi. Colleghi

Anne Alexander e un altro professore o ricercatore) che hanno instradato Regeni sugli studi in Egitto. Essi non hanno voluto rispondere alle domande del pubblico ministero Sergio Colaiocco,

Mi avvio alla conclusione. In materia di indagine e segreti, sul versante mediorientale si vuole quasi una semiguerra all'Egitto. Non gli diamo i pezzi di ricambio degli aerei che combattono il terrorismo in Libia, Egitto e altrove. Attenzione, attenzione, colleghi che voterete. Il subemendamento 4.100/1 del senatore Tarquinio consente di mantenere un rapporto di alleanza in una posizione che comunque chiede la verità, che ritira l'ambasciatore e che fa tutto quello che volete nei confronti dell'Egitto (e che condivido), ma non con un autolesionismo nel disarmare qualcuno che combatte il terrorismo.

che sono depositate presso i Servizi di sicurezza. Le abbiamo lette nell'esercizio delle nostre funzioni parlamentari, con il vincolo della segretezza; quindi ovviamente non dirò cosa c'è scritto. Altri colleghi che le hanno viste hanno interpretazioni diverse dalle nostre. Noi chiediamo però trasparenza, oltre che sul caso Regeni giustamente ai professori di Cambridge

sono passati trentasei anni; francamente, mi pare che sia una era intera. I protagonisti del tempo - ahimè - credo che siano tutti morti o comunque sono fuori dai circuiti istituzionali. Noi vogliamo un po' di chiarezza sul terrorismo; e da quelle carte si capiscono molte cose sul Medio Oriente e su contesti che sono strettamente connessi alla lotta

Vogliamo la verità sul caso Regeni, ma evitiamo di fare il gioco del terrorismo, disarmando chi lo combatte. Io il ritorno dei Fratelli musulmani in Egitto non lo considererei un fatto positivo.

sull'emendamento 4.200, piuttosto che rivolgermi ai relatori e al Governo, preferisco rivolgermi ai cittadini che stanno fuori, perché bisogna fare chiarezza. Cominciamo a leggerlo: leggerlo: «È autorizzata, per l'anno 2016, la cessione alla Repubblica federale di Somalia, a titolo gratuito,» - che poi gratuito non è, vi spiegherò - «di quattro autovetture munite di sistemi di monitoraggio e tracciamento delle reti di telefonia mobile GSM/GPRS (GA 900), nonché di sedici strumenti musicali per banda».

5 Stelle quali: «strumenti musicali». Signor Presidente, cittadini fuori, è inaccettabile che si possa continuare con questo sistema di regalie. Tra le altre

«Si trovano qui in Italia, venite a prenderveli». Perché noi paghiamo il trasporto e le assicurazioni. Tutto questo sistema va ad alimentare i miliardi di euro che da anni diamo in queste missioni internazionali; per l'esattezza, in questo caso si tratta di 1,3 miliardi di euro.

L'articolo 11 della Costituzione è chiaro, non per me, ma per tutti: «L'Italia ripudia la guerra», e dobbiamo assolutamente evitare di armare qualsiasi tipo di popolazione in giro per il mondo. Non va assolutamente bene il discorso di contrasto a

a questa cessione di armamenti, come a tutte le altre cessioni. Davanti a questa cosa dico: ma tutti quelli che hanno fatto le marce per la pace, i pseudosinistroidi all'interno di questo Parlamento, dove stanno all'interno del PD? SANTANGELO *(M5S)*. Uscite fuori davanti a una cosa semplice. Su emendamenti che sono una gran porcata potete semplicemente pigiare il tasto rosso e votare no.

intervengo su questo emendamento, al di là delle considerazioni testé ascoltate, anche per un fatto di equilibrio di copertura finanziaria dell'intero provvedimento. Questo emendamento entrerebbe a far parte del corpo dell'articolo 4, il quale, assieme agli articoli 1, 2 e 3,

è vero che il Governo, soprattutto sul comma 4, ha tenuto anche a specificare il valore dei singoli beni che andava cedendo. Quindi, a mio giudizio,

tramite procedure previste all'interno delle Forze armate, ogni anno considera non più aventi valore strumentale o valore economico. Mi spiego meglio.

andare a esibirsi in queste minuzie, che suscitano anche la giusta protesta di molti colleghi posti dinanzi a una evidenza così risibile o anche camuffata,

a delle dazioni di materiale bellico o anche di supporto civile alle popolazioni.

una facoltà operativa al Governo, che molto spesso opera anche nell'ambito dell'osservanza di trattati. Siamo stati tutti interessati in passato all'osservanza dei trattati con i Paesi frontalieri dell'Africa, per quanto riguarda appunto il contrasto ai fenomeni migratori, e sappiamo benissimo che questi trattati contengono, su richiesta dei nostri interlocutori, per lo più dazioni di materiale, ancor più che dazioni di denaro. Su questo, devo dire di essere molto perplesso per il modo di operare del Governo; molto perplesso di come si voglia costringere il Parlamento, anche attraverso una discussione che molto spesso non può essere approfondita più di tanto, a entrare nel merito di questioni in cui il Parlamento non dovrebbe entrare.

solamente da una determinata ditta che costruisce armi e quindi è una tipologia assolutamente specifica,

il Governo a intervenire con maggiore puntualità. Sugli strumenti musicali a questo punto bisognerebbe anche sapere se siano Steinway o di altra marca. Chiedo scusa ai colleghi per il tempo

il Governo ha fornito, insieme agli emendamenti, le specifiche relazioni tecniche in modo da mettere la Commissione bilancio nelle condizioni di poter apprezzare se vi fossero o meno costi aggiuntivi. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a un emendamento come questo, dove, come si può notare, non c'è alcun impegno di spesa e alcun riferimento a una questione tecnico-finanziaria, nell'ambito della relazione tecnica di accompagnamento è specificato

e l'imballaggio del materiale comporta degli oneri, in questo caso, invece, il Paese terzo richiamato, che è la Somalia, provvederà in proprio a prendere tutti i materiali,

In relazione alla richiesta di portare all'attenzione del Parlamento determinate cessioni, evidentemente questo non è altro che il combinato disposto di due elementi: uno di natura burocratico-amministrativa di carico e scarico e l'altro perché siamo all'interno di cessioni di materiale a un Paese terzo che in genere vengono ratificate dal Parlamento.

e stile la dignità di questo Palazzo. Infatti, se siamo costretti a votare una legge per dare 16 strumenti musicali ad un altro Paese è chiaro che chi legge questa norma domani si

considerato "quello che sta a Palazzo Madama" per votare la consegna di 16 strumenti musicali. Non è una questione di copertura, vale a dire del costo dei 16 strumenti musicali. Chiunque di noi abbia assolto al servizio militare sa che la consegna di 16 strumenti musicali è affidata normalmente

approfitta delle distrazioni dei rappresentanti del Governo, l'Esecutivo

in modo tale che se qualcuno in una trasmissione televisiva dovesse dire che il Senato è inutile io manderò un messaggio per dire che è inutile perché il Governo ci fa votare queste cose.

Si fa per via amministrativa. Se è parte di un accordo, approviamo l'accordo al cui interno ci sono 50 pagine, 100 commi e 200 articoli. Quindi o l'emendamento verrà ritirato o il mio voto sarà contrario. il mio voto sarà contrario. La pallina rossa aveva bisogno, presidente Zanda, di una specificazione. La pallina rossa di Sposetti ha bisogno di questa specificazione.

fatta. Pertanto, proprio perché è un'inezia, fa scaturire delle reazioni, tra cui quella condivisibilissima del collega Sposetti. si potrebbe anche dire «lasciamo correre», perché in questo caso si parla di cedere gratuitamente alla Somalia quattro autoveicoli attrezzati per il monitoraggio di reti telefoniche Noi non lo possiamo neanche sapere: probabilmente lì esiste una nostra banda che ha deciso di tornare senza strumenti donandoli alla banda nazionale di quel Paese. Se però ci vogliamo concentrare sulle dovremmo guardare, ad esempio, quella fatta all'Uganda perché tre elicotteri A109 sono un impegno finanziario non da poco.

forse anche più intelligente. di vestiario, impermeabili da libera uscita (probabilmente saranno quelli in livrea, quelli da festa), che verranno ceduti e lasciati in Libano.

chi ha provveduto a fare la commessa per il rifornimento di 10.000 capi di vestiario per meno di 1.000 uomini

privatistico: se il responsabile abbigliamento della Standa a fine stagione avesse una giacenza di 10.000 capi di vestiario,

Santangelo, che, insieme ad altri suoi colleghi, con l'emendamento 4.2 ha proposto addirittura cessioni di equipaggiamenti e di armamenti all'Afghanistan, a Gibuti, alla Repubblica tunisina, all'Iraq e ad altri.

eventualmente, in un'altra occasione, perché nel contesto del decreto missioni è talmente irrilevante che non vorrei si sprecasse tutto il ragionamento nell'insieme. Proporrei quindi al Governo, che lo ha presentato

che non siano autorizzate cessioni a titolo gratuito di armi e sistemi di armamento a beneficio di Paesi le cui leggi e Governi violano i diritti umani o addestrano e utilizzano manovre di combattimento.

Vorrei dire però che l'attribuzione di falso al relatore da parte del collega Marton, potrei replicarla con un'accusa di falso al senatore Santangelo. Quando infatti il senatore Santangelo ha protestato contro l'emendamento 4.200 delle Commissioni riunite ha esplicitamente fatto riferimento alla circostanza secondo cui in questo emendamento si sarebbe autorizzata la cessione a titolo gratuito alla Somalia di armamenti. Questo è falso. È falso, perché l'emendamento prevede, oltre ai famosi strumenti musicali, la cessione di quattro autovetture munite di sistema di monitoraggio e tracciamento delle reti di telefonia mobile, che sono quelle adoperate dalle nostre forze di polizia anche per le intercettazioni per le intercettazioni telefoniche e ambientali.

non si trattava né nell'emendamento 4.2 del Movimento 5 Stelle, né nell'emendamento 4.200 delle Commissioni riunite. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questa è la verità, poi si è deciso di ritirare l'emendamento, ma almeno ristabiliamo, anche per una correttezza nei confronti dei cittadini a cui il senatore Santangelo si è rivolto e che non hanno il fascicolo degli emendamenti davanti, la verità dei fatti.

non credo che facciamo un buon servizio prendendo spunto da elementi che possono avere anche un carattere pittoresco, come i tromboni, per arrivare alla soppressione e al ritiro di emendamenti o di parti del provvedimento in esame, che per noi possono essere anche insignificanti

ci provo anche perché il tema è piuttosto delicato. Sono trascorsi sette anni da quel tragico 29 giugno 2009 in in cui il treno merci 50325 deragliò nella stazione di Viareggio e la fuoriuscita di gas da una cisterna continente GPL provocò un disastro ferroviario senza precedenti. Morirono ben 32 persone e un gran numero di feriti di allora sono ancora oggi sottoposti a cure mediche pesanti. La procura di Lucca ha rinviato a giudizio 42 imputati, 33 persone fisiche e nove società. I capi di importazione sono: disastro ferroviario colposo, incendio colposo, omicidio e lesioni colpose plurime, oltre a numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La sentenza di primo grado sarà emessa prima del termine di prescrizione imminente (fine 2016), ma questi reati saranno prescritti prima della sentenza di appello. I familiari con le loro forze stanno lottando perché sia fatta giustizia e la prescrizione sarebbe un ulteriore grande insopportabile dolore. Poiché il processo si è caratterizzato per una situazione di grave squilibrio tra diritti delle persone offese e diritti degli imputati, avendo le Ferrovie dello Stato mobilitato per difendere i dirigenti imputati e le sue imprese ben 25 avvocati di chiara fama, oltre alla schiera di assistenti di ciascun avvocato, ho presentato un'interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti per sapere chi sta pagando le ingentissime spese dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato, società al 100 per cento di proprietà dello Stato. Oggi la città di Viareggio ricorda i morti di quella notte maledetta per stringersi intorno ai familiari delle vittime e ribadire la necessità di giustizia che, anche oggi, a distanza di sette anni, non è arrivata e rischia di non arrivare mai se scatterà il meccanismo trappola della prescrizione per il quale, dal secondo grado in poi, spariranno incendio e lesioni colpose come se niente fosse accaduto. Voglio ringraziare la Commissione infortuni sul lavoro per avere deciso di proiettare a settembre il video «Ovunque Proteggi», che sta facendo il giro del mondo e che è stato premiato a Cannes perché riesce, nello spazio di un cortometraggio, a narrare con grande efficacia il carico di dolore di un'intera città ferita che grida: «No alla prescrizione e sì alla giustizia e alla sicurezza». *(M5S)*. Signor Presidente, il tema è sempre lo stesso. Ovviamente è una giornata di lutto per tutti noi. È l'anniversario della strage della stazione di Viareggio, ormai il settimo. Ricordo a tutti che quella strage provocò 32 vittime: perirono donne, uomini e bambini. Purtroppo, oggi persiste il rischio di prescrizione per alcuni reati, quali l'incendio e le lesioni colpose,

Se una cisterna carica di GPL deragliò ed esplose, portandosi via la vita di 32 persone, qualcosa non funzionò. Le persone morirono straziate dal fuoco e dalle fiamme, anche dopo molti giorni di terribile agonia. L'allora amministratore delegato Moretti, solo undici mesi dopo quella immane tragedia, per la quale è imputato insieme ad altre 32 persone, fu onorato con il titolo di cavaliere del lavoro dall'ex presidente Giorgio Napolitano, onorificenza che dovrebbe essere attribuita a chi è un esempio per tutti i cittadini. Mai onorificenza fu peggio conferita, soprattutto se ricordiamo che durante la gestione dell'ingegner Moretti ci furono quasi 50 morti tra macchinisti e addetti alla manutenzione, dipendenti delle Ferrovie e di ditte appaltatrici, cui si aggiungono più di 60 passeggeri morti per incidenti ferroviari, spesso causati da gravi carenze e mancati investimenti nella sicurezza. Penso che la politica non debba restare indifferente all'appello lanciato dalle associazioni dei familiari delle vittime, che chiedono da molti anni che venga revocato il titolo di cavaliere del lavoro all'ingegner Moretti. Già dal 19 febbraio 2014, a nome del Movimento 5 Stelle, presentai una mozione per la revoca del titolo di cavaliere del lavoro, ma da allora giace nei cassetti.

tutti i senatori (in particolar modo toscani), sicura che non sarebbe mancata la condivisone e la sottoscrizione della mozione. In questi giorni le associazioni coinvolte hanno ricevuto il sostegno ad una carta d'intenti sottoscritta da molte amministrazioni comunali, provinciali e dalla Regione, in segno di solidarietà: a ulteriore convincimento, ora più che mai, che bisogna dare un segnale forte e chiaro, pena la perdita di credibilità. Riusciremo tutti insieme a fare una battaglia di giustizia, onore e verità? Per la cronaca, ricordo che fu Matteo Renzi a incaricare Moretti, da amministratore delegato delle Ferrovie a amministratore delegato di Finmeccanica, con conseguenti straordinari vantaggi economici e di carriera. Riuscirà questo Senato a remare contro la volontà di re Giorgio Napolitano? Lo vedremo a breve. Basta pacche sulle spalle. I cittadini e i familiari delle vittime vogliono i fatti.

Presidente, chiedo di prestare attenzione alla tragedia che si sta consumando in Calabria, esattamente nella Piana di Gioia Tauro, con riferimento al porto di Gioia Tauro, che doveva rappresentare un fiore all'occhiello della Regione per poter permettere alla stessa di riprendere quota in termini economici, sociali e industriali nell'area mediterranea, per poter permettere ai calabresi di non dovere essere costretti - come se vi fosse un destino cinico e baro, come amava dire qualcuno - all'emigrazione. Ebbene, quel porto sta morendo

tra l'altro, pure lui calabrese - del sottosegretario Antonio Gentile. In sostanza, 442 lavoratori temono che a breve possa concludersi un'esperienza che doveva essere risolutiva. Di fatto, invece, per la l'ignavia di istituzioni politiche, che dovrebbero tutelare il territorio in maniera sana, essi sono stati abbandonati a loro stessi con un operatore che fa quanto

in questo campo sono i cinesi coloro che stanno spostando le direttrici commerciali verso l'Adriatico, il porto di Gioia Tauro, che - torno a ripetere - doveva essere una speranza, adesso è morto. Desidero concludere il mio intervento ricordando a tutti che per quanto nel 2015 il PIL del Sud sia cresciuto dell'1

Questo significa che la Calabria, ancora più delle altre Regioni, sta diventando un luogo da cui è necessario andare via ed emigrare. Vi ricordo che il tasso di occupazione in Italia è pari al 56,3 per cento, mentre in Calabria al 38,9 anche la Calabria faccia parte dell'Italia e il Governo se ne dovrà ricordare visto che tale Regione è essa stessa molto spesso inconsapevole dei suoi doveri. Ricordo ancora che circa due terzi dei disoccupati calabresi sono disoccupati di lungo corso.

entrate secondarie e chiudersi in prefetture nelle quali è solennemente difeso come i simulacri del potere che non hanno nulla di democratico.